che il ministro Amato, che evidentemente abita in un altro Paese e si accorge del problema immigratorio solo quando vede le trasmissioni di Santoro in televisione, venga al più presto in Aula a riferire sulla reale situazione di sicurezza dei cittadini italiani.

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo per schede, secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 1, del Regolamento. Ciascun senatore riceverà una scheda sulla quale potrà indicare tre nominativi riferiti alla elezione dei componenti effettivi e tre nominativi riferiti alla elezione dei componenti supplenti. Per le operazioni di voto è stata predisposta un'urna. Dopo che avranno votato i senatori presenti in Aula al momento dell'effettuazione della chiama, l'urna resterà aperta per dare modo agli altri senatori di partecipare alla votazione. I senatori, chiamati in ordine alfabetico, passeranno sotto al banco della Presidenza e deporranno la scheda nell'urna predisposta.

Allegrini, Allocca, Amati,

Battaglia Antonio, Battaglia Giovanni, Bellini,

Binetti, Biondi, Bobba, Boccia Antonio, Boccia Maria Luisa, Bodini,

Bulgarelli, Burani Procaccini, Butti,

Colombo Furio, Comincioli,

Cossutta, Cursi, Curto, Cusumano,

Di Bartolomeo, Di Lello Finuoli, Dini,

Ferrante, Ferrara, Filippi, Finocchiaro, Firrarello,

Firrarello, Fisichella, Fluttero, Follini, Fontana, Formisano, Forte,

Giaretta, Girfatti, Giuliano, Gramazio, Grassi, Grillo,

Lusi* *Maccanico, Maffioli, Magistrelli,

Manzella, Manzione, Marconi,

Martone, Massa, Massidda,

Mazzarello, Mele, Menardi, Mercatali, Micheloni, Molinari, Monacelli, Mongiello,

Morando, Morgando, Morra,

Pastore, Pecoraro Scanio, Pegorer, Pellegatta,

Pittelli, Poli, Polito, Pollastri,

Ramponi, Randazzo, Ranieri, Ripamonti,

Roilo, Ronchi, Rossa,

Tibaldi, Tofani, Tomassini, Tonini,

Turigliatto* *Valditara, Valentino, Valpiana, Vano, Vegas,

Vizzini. *Zanda, Zanettin, Zanoletti, Zanone, Zavoli,

Ziccone, Zuccherini.*

vorrei sottoporre all'attenzione sua e dei colleghi un problema che mi sembra di una certa importanza. Il presupposto di fatto è il seguente: avevo presentato un'interrogazione parlamentare chiedendo al Governo notizie in ordine al cosiddetto emendamento Fuda, alla quale è stata data risposta in Commissione. Il Governo, nel rispondere a una specifica domanda che riguardava l'elenco delle persone che si sarebbero eventualmente avvantaggiate da tale emendamento, ha fatto fatto rinvio a un elenco di nomi trasmesso dalla Corte dei conti, richiamando ragioni di *privacy*. In ragione della risposta del Governo, il presidente Bianco ha disposto che si potesse consultare l'elenco stesso, ma che non se ne potesse estrarre copia. La posizione del presidente Bianco è stata oggetto di discussione in Commissione sia i componenti della maggioranza sia i componenti dell'opposizione hanno manifestato forti dubbi in ordine alla legittimità del percorso da lui scelto. Devo altresì dare atto al presidente Bianco che, nella lettera con la quale ha investito la Presidenza della risoluzione del problema, si è fatto carico di rappresentare l'andamento dei fatti e la presenza di forti dubbi in Commissione, che riguardavano - ripeto - sia la maggioranza sia l'opposizione. Orbene, oggi il presidente Bianco ha dato lettura della sua risposta, presidente Marini, in Commissione. Nella sostanza, lei, in questa risposta, dice che è chiaro che la *privacy* non può essere opposta a ragioni di preminente interesse pubblico, come sono quelle tipiche della funzione parlamentare e in particolare del sindacato ispettivo, ha altresì affermato che, nel bilanciamento tra l'interesse alla *privacy* e l'interesse pubblico, sono possibili forme diverse di consultazione. Orbene, Presidente, io vorrei adesso liberare il campo dal problema emendamento Fuda ed elenco dei soggetti sottoposti a procedimento contabile

ci troviamo di fronte ad un elenco di oltre 3.800 nomi (siamo in presenza di circa 300 pagine di nominativi, di importi contabili, di procedimenti), che evidentemente non possono

rappresentato nella sua lettera; quello che voglio dire io è che nel bilanciamento tra l'esigenza della *privacy* e quelle proprie del sindacato ispettivo,

con riferimento ad una norma sbagliata, tanto sbagliata che voi stessi avete ritenuto di doverla vanificare attraverso un decreto-legge che poi è stato convertito in legge, una norma che ha dato vita ad un forte dibattito in queste Aule e che ha creato anche un certo tipo di allarme nel Paese, in ragione dell'entità dei recuperi contabili che sarebbero venuti meno proprio a seguito di quell'emendamento. In altri termini, signor Presidente, noi vogliamo semplicemente capire qual era la portata di quell'emendamento, ma le modalità di consultazione da lei indicate non ci consentono tale verifica e sostanzialmente vanificano il sindacato ispettivo, che è una delle prerogative dei parlamentari.

volessimo farlo. L'effetto di questa decisione è dunque solo di rendere più difficile l'esercizio di una funzione costituzionalmente protetta e rilevante: la funzione ispettiva del parlamentare, che è fondamentale nel sistema democratico. Penso, signor Presidente, che si possa correttamente chiedere al parlamentare di mantenere la riservatezza, ma non si può opporre la riservatezza al parlamentare nell'esercizio della funzione ispettiva. Intanto,

e questo già è un dato che lascia intendere che ci sia un problema di funzionamento del sistema democratico. Aggiungo che, nella specie, si tratta - come ricordava il collega Palma - di un elenco che aveva a che fare con la nota vicenda della della sanatoria davanti alla Corte dei conti; quindi, per definizione, siamo in una materia che attiene all'uso del denaro pubblico. In quell'elenco possono essere presenti solo persone che hanno gestito denaro pubblico o che hanno ricoperto hanno ricoperto cariche di gestione e di governo e il fatto che abbiano o meno arrecato danno erariale è ovviamente un elemento rilevante ai fini della giusta valutazione dell'opinione pubblica nei loro confronti. Questo aggiunge motivazioni al fatto che non si dovesse porre ostacolo di alcun genere al pieno esercizio della funzione ispettiva. Ritengo la decisione della Presidenza dell'Assemblea sbagliata, ritengo che dovrebbe essere modificata; sarebbe assai sgradevole se si dovesse arrivare a questo effetto modificando la legge sulla *privacy*, in modo tale da far sì che non si possa da quella normativa trarre elementi di opposizione e di contrasto

Il senatore Palma ha riferito bene la questione, così com'è: noi ci siamo trovati dinanzi all'interrogazione e al Governo che ha fornito alla Commissione affari costituzionali un elenco di 3.800

nell'Aula del Senato il decreto-legge n. 23, che reca disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, dopo l'esame dell'altro ramo del Parlamento, nel corso del quale sono state apportate significative modifiche. Ricordo anche che il decreto dovrà essere convertito entro il prossimo 19 maggio a pena di decadenza dello stesso. Entrando nel merito, rispetto al testo licenziato in quest'Aula in prima lettura, la principale novità è costituita dalla riformulazione dell'articolo 1-*bis*, introdotto in Senato, volta ad azzerare la quota fissa sulla ricetta riguardante le prestazioni di specialistica ambulatoriale. In proposito, si tratta di una modifica in linea con l'orientamento emerso già in prima lettura quando, si ricorderà, tale quota - introdotta all'articolo 1, comma 796, lettera della legge finanziaria per il 2007 - era stata sensibilmente ridotta, passando da 10 a 3,5 euro. A conferma dell'impegno politico del Senato in questa direzione, si rammenta altresì che nel corso dell'esame sia della legge finanziaria che, successivamente, del decreto- legge n. 300 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 2007, era stato presentato più di un emendamento soppressivo o volto a limitare la vigenza delle citate disposizioni in materia di *ticket*. In particolare, con la legge n. 17 del 2007 la vigenza di tali disposizioni era stata limitata alla data del 31 marzo, ovvero all'entrata in vigore di misure alternative che avessero effetto equivalente sotto il profilo finanziario e che dovevano in quel caso essere stabilite a livello regionale. Nel corso dell'esame del testo del presente decreto-legge, così come licenziato in prima lettura dal Senato, la Camera ha incrementato la copertura economica, ora pari a 511 milioni di euro per il 2007 (rispetto ai 350 milioni di euro previsti nel testo accolto dal Senato), modificando nel contempo anche le riduzioni delle autorizzazioni di spesa interessate, in conformità all'impegno assunto dal Governo nel corso della discussione al Senato. Su tale argomento interverrà il relatore Tecce. La soppressione del *ticket* sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale anche per gli assistiti non esenti e l'individuazione di una copertura finanziaria adeguata, rappresentano oggi una conferma della maggiore attenzione da parte di questa istituzione nei confronti delle politiche sociali. È stata anche soppressa la norma che avrebbe consentito di bloccare per un anno le azioni esecutive riguardanti i debiti sanitari nei confronti delle aziende creditrici del sistema sanitario nazionale site nelle Regioni interessate dal ripiano finanziario. Si segnala che la Camera ha introdotto ulteriori modifiche all'articolo 1 dirette a rafforzare la trasparenza, ma anche il controllo e la verifica degli adempimenti previsti in tema di rientro dai disavanzi. In particolare, si prevede che il Ministro dell'economia debba trasmettere gli esiti della verifica annuale dei piani di rientro al presidente della Corte dei conti, anche al fine di avviare un eventuale giudizio di responsabilità. Inoltre, si dispone che il decreto ministeriale di ripartizione dell'importo stanziato (3 miliardi di euro) a titolo di regolazione debitoria, sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato. Infine, sempre a tale riguardo, si sancisce che il Ministro dell'economia, sentito il Ministro della salute, trasmetta una relazione sullo stato del monitoraggio e del riscontro dell'estinzione dei debiti. Nel corso dell'esame in Commissione sono stati presentati diversi emendamenti che si possono far risalire a tre sostanziali obiettivi: quello di introdurre sanzioni o automatismi in ordine al mancato rispetto dei piani di rientro; quello di modificare la copertura di spesa; quello di inserire la Conferenza Stato-Regioni tra gli organi competenti ad esprimere un parere sul monitoraggio e sul riscontro dell'estinzione dei debiti. Tali emendamenti (che oggi vengono ripresentati in Aula) sono stati respinti ad eccezione di due,

al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo - lo sottolineo - 2001-2005, nei confronti di quelle Regioni che hanno già sottoscritto con lo Stato un accordo per i piani di rientro (il cosiddetto patto per la salute), accedono al fondo transitorio, già previsto dalla legge finanziaria 2007 e adottano specifiche misure fiscali per la copertura dei disavanzi o destinano al settore sanitario quote di entrate derivanti da misure fiscali già adottate o quote di tributi erariali attribuite alle Regioni. A tal fine (questo è l'aspetto dal punto di vista del bilancio) è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria (come sottolineava la collega Emprin Gilardini), la spesa di 3 miliardi di euro per il 2007, che verrà ripartita tra le Regioni interessate secondo quanto concordato nel Patto, anche in sede di Conferenza Stato-Città-Regioni. Nel corso dell'*iter* del disegno di legge di conversione del decreto in esame, il Senato, in prima lettura, aveva disposto - ne ha già parlato in termini di valore politico come diritto alla salute - la riduzione da 10 a 3,5 euro, limitatamente al 2007,

L'importo atteso dalla misura, quantificato dalla legge finanziaria in 811 milioni di euro nel 2007, risultava quindi rideterminato in 461 milioni di euro, visto il periodo dell'anno che andava a coprire; corrispondentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre lo Stato, veniva incrementato, sempre per il 2007, di un importo pari alle minori entrate, ossia 350 milioni di euro. Dico questo perché ho il dovere, come relatore, di informare soprattutto circa le modifiche intervenute alla Camera dei deputati. Per quanto concerne i profili di copertura, il comma 2, introdotto al Senato, autorizzava appunto la spesa di 350 milioni di euro al cui onere si provvedeva mediante la riduzione di diversi fondi, quali il Fondo per i Paesi in via di sviluppo, il Fondo per la famiglia, il Fondo per le autosufficienze (tema sul quale c'è stata una discussione vivace in quest'Aula). Tuttavia, nel corso dell'esame alla Camera, questa modalità di copertura ha suscitato perplessità e critiche sia da parte dell'opposizione che della maggioranza, in conseguenza del fatto che si sarebbe andato ad incidere, in percentuale notevole, su fondi creati o implementati proprio con la legge finanziaria per il 2007. Non è sembrato accettabile, soprattutto, che fossero intaccate risorse destinate a politiche sociali rilevanti e di qualità. Nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite bilancio e affari sociali della Camera, è stato approvato un emendamento con il quale si dispone la totale eliminazione della quota fissa, ovvero dei *ticket*, sulle ricette relative a prestazioni sanitarie per l'anno 2007 e si provvede alla copertura della spesa necessaria, pari a questo punto a 511 milioni di euro (perché vi è eliminazione totale nel periodo dell'anno conseguente) per il 2007, nel seguente modo: 100 milioni mediante riduzione del Fondo per i debiti pregressi e 411 milioni mediante l'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per le politiche comunitarie (tale fondo era stata la prima proposta di copertura all'emendamento, poi cambiata successivamente in discussione in Commissione bilancio al Senato). Su tale emendamento, il Governo si è espresso favorevolmente garantendo, altresì, che al reintegro dei fondi si provvederà con idoneo provvedimento subito dopo l'assestamento del bilancio. Ricordo inoltre che sulla proposta allora formulata dal Governo, relativa all'utilizzo del fondo di rotazione ai fini di copertura della riduzione del *ticket*, il Senato aveva espresso parere contrario manifestando alcuni profili problematici che riguardavano essenzialmente il rischio che tale copertura potesse determinare una dequalificazione della spesa. A fronte di oneri di natura corrente, infatti, si stabiliva l'utilizzo delle risorse del fondo rotativo, che ha natura di conto capitale. Veniva rilevato, inoltre, il rischio che l'utilizzo di quota-parte delle risorse del Fondo per le politiche comunitarie, nella misura indicata, potesse pregiudicare l'attuazione di interventi già finanziati. Su questo aspetto ho il dovere d'informare invece l'Aula del Senato che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in risposta a tale ultima obiezione (il rischio cioè che non si finanziassero politiche comunitarie approvate dal Parlamento), ha rassicurato, sia nel corso dell'esame alla Camera sia ieri intervenendo in Commissione bilancio, precisando che il notevole ritardo ritardo registrato nell'anno in corso nell'approvazione dei programmi comunitari, per i quali è previsto l'utilizzo delle risorse del fondo, consente il parziale utilizzo per questi mesi di quota-parte del fondo stesso, in vista peraltro, come già detto, della reintegrazione dello stesso dopo l'assestamento. Quanto al rischio paventato di una dequalificazione della spesa, si precisa che le modalità indicate dall'emendamento per l'utilizzo parziale delle risorse del fondo, cioè il versamento di tali risorse nello stato di previsione delle entrate, per la successiva riassegnazione al Fondo sanitario nazionale, sembrano idonee ad evitare tale eventualità. Peraltro, in numerose occasioni, anche recenti, il legislatore ha disposto l'utilizzo delle risorse del fondo di rotazione per la copertura di oneri di parte corrente. di oneri di parte corrente. L'attuale livello dei disavanzi nella gestione della sanità da parte delle Regioni è talmente grave da incidere profondamente non solo sulla credibilità delle istituzioni regionali, ma sull'intera pubblica amministrazione,

decisamente volti a cambiare le modalità di gestione e utilizzo delle risorse destinate alla sanità nelle Regioni interessate, attraverso rigide misure di correzione e di controllo, che ne limiteranno fortemente le determinazioni. Vorrei sottolineare, infine,

parlamentari competenti. Tale emendamento, a mio avviso, è molto opportuno e serve anche ad evitare che fondi stanziati per ripianare debiti al 31 dicembre 2005 possano essere utilizzati per spesa corrente. L'obiettivo evidente è quello di obbligare le Regioni ad adottare comportamenti e modalità gestionali orientati all'efficienza dei sistemi sanitari regionali, all'eliminazione degli sprechi, a volte davvero intollerabili, e soprattutto alla capacità di rilanciare il diritto costituzionale alla salute in tutto il Paese.

l'articolo 117 della Costituzione e ora la tutela della salute rientra nelle potestà concorrenti Stato-Regioni. Allo Stato pertanto rimane la fissazione dei livelli essenziali di assistenza, ma compete alle Regioni l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni, nonché il modo per farvi fronte, ossia il modo di reperimento delle risorse. Anche in questo caso, dunque, viene violata palesemente la competenza regionale. Per queste tre motivazioni che ci sembrano fortissime, non capziose e non

spese con la contrazione di debiti. Questo viene ad essere stabilito non soltanto riguardo alle Regioni, perché si dice che l'importo di cui all'articolo 1 viene devoluto alla Regione per la riduzione strutturale del disavanzo nel settore sanitario, ma anche per l'ammortamento del debito accumulato fino al 31 dicembre. viene autorizzata da parte della Regione la contrazione di un debito per la copertura di spese in conto corrente, ma c'è di più: lo Stato interviene, contrariamente a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 119, e rifonda i debiti contratti dalla Regione per la copertura di un debito in conto corrente con un'assunzione di debito a suo carico perché non finisce per elevare il debito dello Stato ma per fare un trasferimento sul debito contratto alle Regioni, e quindi in apertissima violazione Ma c'è un'altra cosa che rileva in maniera forte, alla quale poco ci si è appuntati in questo ramo del Parlamento perché riguarda non tanto l'articolo 1, comma comma 1-*bis*, come è stato introdotto e corretto nella copertura nell'altro ramo del Parlamento, bensì il comma 2. Vede, Presidente, il comma 2 ha scarsissima rilevanza ai fini generali e per quanto attiene alla spesa,

le regioni che, con delibera di Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione entro il 27 marzo del 2007...», eccetera, eccetera. Ma cosa significa «27 marzo 2007»? Perché si parla di delibera della Giunta? Sappiamo che la Costituzione dispone che le leggi abbiano carattere universale e quindi siano disposizioni di carattere generale.

Cosa succede e perché ha una rilevanza ai fini della legge di contabilità e quindi ai fini dell'articolo 119 della Costituzione? Perché un'interpretazione *stricto iure* della legge darebbe la possibilità alla Regione Campania di

che considero assolutamente plausibile, accreditata in ambienti giuridici e, per le vie brevi, confortata dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia - darebbe la possibilità ad una sola Regione,

accingo a motivare. Riteniamo che, in realtà, il provvedimento non violi il principio di uguaglianza: l'articolo 3 della Costituzione non fa riferimento alle Regioni ma, appunto,

in grado, una volta ripianati, di rispondere alla capacità di spesa per quanto riguarda i servizi sanitari da offrire, non più impegnati quindi nei pagamenti

l'approvazione, misure di rientro obbligatorie laddove non riescano a rientrare dal disavanzo. È quindi evidente che hanno bisogno di programmare al più presto le eventuali misure di rientro e, comunque, entro l'approvazione dei prossimi bilanci regionali. Infine, per quanto riguarda la terza motivazione

determini i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. È per noi quindi determinante, appunto, la condizione finanziaria, affinché sia poi per le Regioni, intervenire nel dettaglio sull'organizzazione e l'erogazione di tali servizi essenziali di assistenza. È dunque pregiudiziale permettere alle Regioni di avere quell'equilibrio di bilancio senza il quale l'intervento di dettaglio sull'organizzazione e l'erogazione di dei servizi essenziali non potrà essere possibile.

per ricetta sulle prestazioni sanitarie specialistiche, in linea peraltro con quanto già proposto in Senato dalla Lega Nord, permane comunque la nostra contrarietà al provvedimento in esame, che rappresenta una palese violazione del principio di autonomia e responsabilità di ciascuna Regione

vi richiamo ad una maggiore attenzione, innanzitutto per rispetto di chi parla, cioè di noi stessi.

Tale principio, che è alla base della stessa stipula dei «patti di stabilità» sanitari tra lo Stato e le Regioni, trova un esplicito riconoscimento legislativo nel decreto-legge n. 347 del 2001, che sancisce la responsabilità delle Regioni sulla copertura degli eventuali disavanzi di gestione nel settore sanitario. Tale principio, cui il decreto in esame esplicitamente deroga, rappresenta una sorta di criterio fondamentale di riferimento che non può essere reiteratamente disapplicato, pena lo stravolgimento del complessivo equilibrio dei rapporti Stato-Regioni nel settore sanitario. È inoltre politicamente inaccettabile che l'accesso ai 3 miliardi di euro disponibili sia stato riservato solo ad alcune Regioni, quelle meno virtuose, mentre le altre Regioni, non avendo cumulato disavanzi o avendo provveduto tempestivamente con risorse proprie al ripiano dei medesimi, si vedono doppiamente danneggiate dal provvedimento in titolo. Emerge poi il dubbio che i criteri di riparto, indicati nel comma 2 dell'articolo 1, siano stati «studiati a tavolino» al fine di garantire alla Regione Lazio una quota di risorse statali pari addirittura a 2,3 miliardi di euro (quindi circa il 70 per cento delle risorse complessivamente disponibili): si evidenzia, infatti, che il piano di rientro che la Regione ha stipulato con il Governo già prevede di coprire altri 2,3 miliardi di disavanzo, con il ricorso a «provvedimenti legislativi nazionali». È, tuttavia, evidente che un Governo non potrebbe legittimamente approvare un piano di rientro regionale che si affida, per la copertura di una parte ingente del disavanzo, ad un provvedimento che deve ancora compiere il suo *iter* in Parlamento. Per tutte queste ragioni, chiederemo di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1411-B e, su questa richiesta, chiederemo il voto elettronico.

pone le Regioni, che in questi anni hanno elaborato politiche di rigore nel contenimento della spesa sanitaria, nella situazione di vedere sostanzialmente i loro sforzi rispetto all'approccio tenuto da altre Regioni che, di fronte ad una situazione critica di disavanzo, non hanno assunto quei provvedimenti necessari a raggiungere il contenimento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo il primo sofferto passaggio al Senato di questo decreto-legge per il ripiano dei disavanzi pregressi nel settore sanitario e dopo la diciassettesima fiducia posta alla Camera in un anno, ci accingiamo quest'oggi, prevedibilmente, a siglare il terzo e ultimo atto di una storia non bella e tanto meno edificante, scritta dal Governo e da questo Parlamento. È difficile per chi, come noi dell'UDC, intende svolgere non un'opposizione di maniera ma un'incalzante battaglia politica nelle aule parlamentari, volta a sfidare il Governo sulle proposte a favore del Paese, rassegnarsi a questa evidente pratica di schizofrenia politica. Nel corso della prima lettura del provvedimento in quest'Aula, chiedemmo a gran voce l'eliminazione del *ticket* sulla diagnostica. Tale abbattimento fu impossibilitato per il vibrante intervento del ministro della salute Livia Turco che, però, poco dopo, rimettendosi all'Aula, si rassegnò, come gesto estremo, alla riduzione del *ticket* da 10 a 3,5 euro. vorrei evidenziare, non al fine di sperticarmi in una stregua difesa sindacale, come, superata la soglia della Camera anziché quella del Senato, un altro Ministro, quello dell'economia, abbia avuto un'altra opinione e, superando la posizione politica del Ministro della salute, abbia invece accolto favorevolmente la proposta di eliminazione del *ticket*, proposta che noi condividiamo. Non c'è un solo soggetto, però, che esca bene da questa vicenda, non il Governo, costretto a ripensamenti postumi per mascherare incapacità e divisioni presenti nella sua maggioranza, stretta tra una sinistra radicale e massimalista e un sedicente centro moderato non completamente affrancato però da logiche di potere ed esercizi clientelari; non lo sono i destinatari del provvedimento, cioè le Regioni che beneficeranno dei ripiani dei bilanci, perché tutto il Paese verrà a conoscenza della loro cattiva amministrazione e della difficoltà che loro stesse avranno per spiegare le ragioni dello sperpero del denaro pubblico. Onorevoli colleghi, dopo quelli previsti dalle leggi finanziarie per il 2006 e il 2007, il provvedimento oggi al nostro esame costituisce il terzo intervento in due anni da parte dello Stato per il ripiano dei disavanzi sanitari regionali, e ciò in deroga all'obbligo per le Regioni di ripianare i disavanzi sanitari con oneri interamente a carico, come previsto della legge n. 405 del 2001. È questo un intervento, vorrei ricordarlo, su cui continuano a gravare pesanti indizi di illegittimità costituzionale. Si conduce una selezione nella selezione, si premiano senza reticenze alcune Regioni rispetto ad altre e si privilegiano particolarmente quelle che si sono mostrate più spendaccione ed incapaci di razionalizzare le spese. È difficile, pur senza fare ricorso alla retrologia, non supporre che la sanità sia stata considerata, da queste stesse Regioni poco virtuose, come un formidabile strumento clientelare usato prioritariamente per governare i dipendenti e i loro voti e non tanto per soddisfare il diritto alla salute da parte dei cittadini. Vorrei capire se, in presenza di una evidente discriminazione, persistente sia tra quelle Regioni che hanno accumulato disavanzi nel periodo 2002-2005 e ammesse al finanziamento, oltre che tra quelle che hanno adottato comportamenti virtuosi, non si violi il principio di eguaglianza, o se possa essere considerato buon andamento della pubblica amministrazione il sanare l'inefficienza di alcune Regioni, disincentivando e demotivando nel contempo le altre che hanno adottato invece comportamenti virtuosi. Onorevoli colleghi, la modifica delle competenze e degli assetti istituzionali, operata con la riforma del Titolo V, attribuisce una più forte assunzione di responsabilità alle Regioni, ma con il presente decreto-legge, invece, lo Stato assurge paradossalmente al ruolo di badante per quelle amministrazioni regionali che hanno prodotto un maggior *deficit* sanitario, sollevandole di fatto da ogni responsabilità e premiandole con il trasferimento di ingenti risorse finanziarie per il ripiano del disavanzo. Certamente la questione dei disavanzi sanitari delle Regioni è una grandezza invariabile del nostro sistema sanitario con la quale anche i precedenti Governi hanno dovuto fare i conti, ma non possiamo dimenticare che, a partire dal 2001, con l'accordo tra Stato e Regioni, il debito dovrebbe essere responsabilità di queste ultime, che possono utilizzare a tal fine strumenti di controllo della spesa sanitaria come la leva fiscale o lo storno di risorse da altri capitoli di bilancio. Dal dettaglio delle risultanze regionali contenuto nelle certificazioni trimestrali prodotte dalle Regioni per l'anno 2005 rileviamo una difformità di comportamenti. A fronte, cioè, di Regioni che hanno puntato sul controllo della spesa o che hanno introdotto maggiorazioni sulle addizionali IRAP e IRPEF, accanto a Regioni che hanno impiegato risorse autonome stornate dal bilancio, ci troviamo alla presenza di Regioni che non hanno adottato alcuna misura di copertura. Resta così il sospetto che i supposti piani di rientro finiscano con l'essere non piani virtuosi, ma semplicemente piani economici che trovano la propria ragione d'essere in tanti, troppi lavori fatti a risparmio o in economia, dai quali, pur con qualche ragionevole dubbio, discendono spiacevoli e a volte drammatiche situazioni, come gli otto decessi dell'ospedale di Castellaneta, dove ai pazienti ricoverati nell'UTIC è stato somministrato perossido di azoto in luogo dell'ossigeno. Il provvedimento rappresenta dunque una violazione del principio di uguaglianza e una grave iniquità nei confronti di quelle Regioni virtuose che hanno saputo gestire in modo oculato la spesa sanitaria, anche attraverso l'introduzione di imposte impopolari, ma necessarie per far fronte ad essa. Sappiamo di certo che i malati sono incolpevoli, ma, signor Presidente, non lo sono quegli amministratori e dirigenti incapaci e irresponsabili, che ancora siedono, visto che nessuno si è accinto a presentare il conto, sulle loro poltrone. La legge prevede, punendo le Regioni che non applicano la disciplina vigente, la decadenza dall'incarico di quegli amministratori responsabili dei dissesti sanitari e l'impossibilità di accedere alle risorse messe a disposizione dallo Stato per il ripiano dei disavanzi. Il Governo, invece, con questo decreto non solo ha pensato bene di non prenderla in considerazione, ma ha addirittura ritenuto di continuare ad affidare il progetto di risanamento della sanità esclusivamente ai malati e ai cittadini, considerati nella fattispecie degli utili bancomat da spennare. Oggi, con i tre miliardi di euro ripianate i debiti, ma continuate a non dire nulla degli appalti, delle esternalizzazioni, degli incarichi, degli stipendi faraonici assegnati ai *manager*, che, diciamocelo chiaro, spesso vantano nei loro *curricula* professionali delle lunghe anticamere trascorse negli uffici degli assessori regionali di turno. Con le ripetute sanatorie, con il cosiddetto mille proroghe per gli enti locali che hanno sforato il Patto di stabilità 2006 e con l'ennesimo stanziamento per l'emergenza rifiuti in Campania non facciamo che continuare ad incentivare i comportamenti irresponsabili. Sono i ripiani dei disavanzi con fondi statali gli atti che generano sperequazioni ingiuste per chi è più virtuoso e che conducono all'irresponsabilità e al mantenimento delle disfunzioni. È necessaria una riforma organica tesa a riorganizzare il settore sanitario, capace di adottare una revisione e una razionalizzazione dei criteri di spesa e, soprattutto, incline ad una maggiore responsabilizzazione delle Regioni, con l'attribuzione di adeguati strumenti finanziari. Quando nell'ultima legge finanziaria il Governo Prodi impose il *ticket*, l'UDC fu contraria, ed oggi, pur di fronte a questa inversione ad U, che salutiamo felicemente, nella traiettoria dei ripensamenti continuiamo a dire che meglio sarebbe stato però utilizzare una piccola parte delle risorse del famoso tesoretto per la completa e definitiva soppressione di questa tassa invisa ai cittadini, per la quale invece si propone un semplice arrivederci a dicembre 2007. Non possiamo non rilevare il balletto di cifre del Governo, che prima mette il *ticket* in finanziaria, poi lo diminuisce al Senato, arriva alla Camera e lo elimina, avvertendo però che si tratta di una sospensione temporanea e solo per il 2007, quindi al Senato lo riconferma e «speriamo che....». Insomma, di tutto e di più, un di più che non genera sicuramente quel necessario clima di fiducia che dovrebbe essere alla base del rapporto cittadino-Stato. In questa confusione abbiamo almeno apprezzato la scelta del Governo di modificare la decisione circa la sospensione delle procedure esecutive e dei pignoramenti. Esistevano profili di incompatibilità rispetto alla disciplina comunitaria in materia di transazioni che avrebbero sicuramente determinato l'attivazione di procedure di infrazione della direttiva n. 35 del 2003, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, producendo conseguentemente riflessi finanziari non previsti in termini di sanzioni e spese. Ad oggi lo Stato rimborsa, in media, dopo un anno, quando i termini di legge sono invece di 150 giorni al massimo. Questa disposizione aveva creato un allarme per le aziende del settore, perché bloccava per un anno i pignoramenti e i decreti ingiuntivi da parte dei creditori del Servizio sanitario nazionale. Secondo la normativa vigente, l'esecutività dei decreti ingiuntivi scatta il centocinquantesimo giorno decorrente dalla notifica del titolo, ed il relativo pagamento (mai per intero) avviene dopo circa due anni, attese le lungaggini dell*'iter* processuale. Quindi, circa tre anni di attesa, che con gli interessi sarebbero diventati quattro. Per avere una dimensione del fenomeno, basterebbe ricordare che la Corte dei conti, in un rapporto del luglio 2006, ha calcolato in 22 miliardi di euro l'esposizione complessiva del sistema sanitario nei confronti dei soli fornitori, cui vanno aggiunti i crediti del 2006 e del 2007. Tale situazione sarebbe diventata insostenibile per molte aziende, che oltretutto avrebbero subito persino l'aumento - ove applicato - delle addizionali IRAP, proprio per sanare i disavanzi sanitari. Ancora una volta si sarebbero penalizzati soggetti estranei ai dissesti e premiati coloro che ne sono stati responsabili. In definitiva, questo provvedimento non può essere votato, è niente altro che un odioso colpo di spugna sulle responsabilità, un atto che assegna ciecamente premi e punizioni e dimentica i veri problemi, quelli che dovrebbero essere prioritariamente affrontati:

nella quale ovviamente i primi dubbiosi erano anche tanti componenti della vostra maggioranza. Non ci scandalizza tanto l'obiettivo di un ripiano, una piaga che è avvenuta in passato e che potrà verificarsi

e punisce quelle che per tempo hanno messo in atto tutti i meccanismi per poter rimanere entro i limiti di spesa concessi. È fortemente discriminatorio, come ricordava il collega senatore Galli, in quanto non consente l'accesso a questi fondi, con pari equità, a tutte le Regioni. È dissennato, perché non pone in maniera idonea i controlli, ed è punitivo per i cittadini. Se infatti, da un lato, si vuol far apparire una mano misericordiosa che aiuta ed accompagna le Regioni inaffidabili sul cammino del ripiano della spesa, dall'altro, consente altri tagli, ulteriori imposizioni fiscali su altre entrate e su altri servizi dei cittadini.

si allunga sempre più e in quella lista di attesa ci si aggrava e si muore; non attacca la lista dei problemi e delle priorità,

soprattutto, non si interessa della sicurezza di cui in questi giorni il Governo e il Ministro si riempiono la bocca, ma della quale ancora in questo Parlamento non è pervenuta una riga scritta, ma solo dichiarazioni d'intenti,

perché, in qualità di Presidente della Commissione d'inchiesta, ho rispetto dell'autorità inquirente e della magistratura e perché in molti casi la Commissione stessa ha deciso di secretare gli atti acquisiti.

lo siamo anche del fatto che quell'elargizione cospicua a Regioni così inaffidabili altro non è che una cambiale inesigibile. Anche in questa lettura abbiamo presentato degli emendamenti e degli ordini del giorno, ma sono poche le illusioni che possiate accoglierli. Quindi, il provvedimento vedrà ancora danneggiati e beffati quelli che sono stati virtuosi e, soprattutto, vedrà puniti i cittadini di quelle Regioni: i più facoltosi saranno obbligati a fare i viaggi della speranza, i più indigenti vedranno approfondire il divario tra loro ed il resto d'Italia e calpestati i loro diritti costituzionali.

costano meno di 10 euro, non avete chiesto una compartecipazione, ma avete lucrato sulla sofferenza della gente. Avete cercato di guadagnare sulle malattie, sui livelli essenziali di assistenza, vale a dire su quelle cure per le quali in tutta Italia dobbiamo dare garanzie. Avete fatto una cosa odiosa ed oggi, dopo le pressioni provenienti non solo dall'opposizione, ma dalla piazza e da quei pochi di voi che hanno avuto la delicatezza di leggere il provvedimento,

esclusivamente a Regioni che, guarda caso, sono quelle che hanno speso di più, che non hanno fatto il benché minimo passo indietro per rientrare di quelle spese, alla faccia di quelle Regioni che, invece, onestamente, con grande difficoltà, avevano già provveduto, dolorosamente, a rientrare dei loro debiti. State dando un assegno in bianco a colui che si è già dimostrato moroso, se non truffatore. Credo che nessun cittadino, neanche un ragazzino, farebbe una cosa del genere. Ecco perché non dovete gloriarvi di questo ed ecco perché non siamo d'accordo. L'unica cosa che ci mette in forte imbarazzo è che ci rendiamo conto che i cittadini di quelle Regioni che hanno questo *gap* non hanno nessuna colpa; la colpa è degli amministratori.

esclusivamente come portafogli da spremere per risolvere i problemi della sanità ed ora state facendo pagare a tutta una Nazione i danni provocati da alcune Regioni che, guarda caso, sono tutte a maggioranza di centro-sinistra. Per concludere,

difettano di tutti quei paletti necessari per garantire che questo prestito non solo ritorni, ma sia finalizzato alla qualità. Di fatto, si tratta di un razionamento, perché voi state chiedendo dei piani di rientro economici sulla qualità del servizio; sulla qualità del servizio sanitario non c'è niente, non c'è nessuna garanzia, ci sono soltanto dei "vorrei", dei condizionali, dei *desiderata*, che naturalmente non sono delle garanzie. Su certi provvedimenti - ha avuto il coraggio qualsiasi Governo di farlo - ci avete criticato nel corso della precedente legislatura perché noi stavamo razionalizzando, nel tentativo di trovare un modo per evitare che ci fosse uno spreco. Voi dite «noi proseguiamo lavoro»; il vostro lavoro ha un'altra parola: non razionalizzare, ma razionare, togliere servizi. Basta guardare i dati, i quali indicano che da quando ci siete voi le liste d'attesa in tutta Italia si stanno moltiplicando. L'altro giorno nella mia città è morta una persona perché perché aveva necessità di fare degli esami; ha dovuto attendere tanto di quel tempo per poter fare una risonanza alla mammella, per un tumore, che ci ha lasciato prima di fare l'esame;

non è un patrimonio solo del centro-destra o del centro-sinistra: è un patrimonio di tutti noi. Allora imparate anche voi, cari colleghi. Qualche volta anch'io sono distratto di fronte a certi provvedimenti, ma quello in esame è molto importante;

anni a venire (ammesso che duriate tanto per poter avere i ritorni, perché credo che la piazza stia dicendo qualcosa di ben preciso); siccome questo provvedimento che state portando avanti pretende ma con il condizionale - che ci sia un ritorno, che le Regioni diano conto delle spese sostenute e di come sono intervenute anche per porre dei limiti, noi vigileremo, vi controlleremo e interverremo. Spero che voi abbiate l'onestà almeno di ammettere che avete sbagliato a danno dei cittadini.

Presidente, colleghi, vedendo il provvedimento che torna dalla Camera dei deputati così com'è stato modificato, debbo sinceramente plaudire - e con me penso lo faccia tutta l'Aula del Senato - al fatto che ancora vige, in maniera seria dal punto di vista costituzionale, il nostro sistema bicamerale. Per fortuna, come diceva il collega Gramazio, esiste il sistema bicamerale, che ci ha consentito - parlo come opposizione - di raggiungere quei risultati che inutilmente avevamo tentato di far capire alla maggioranza e al Governo erano quelli che pensavamo logici. Mi riferisco, in particolare, agli emendamenti che sono stati poi approvati dalla Camera e che hanno portato all'abolizione dei *ticket*. Vorrei ricordare che, come Gruppo di opposizione, presentammo

e che la Camera ha giustamente tolto. Quindi, plaudiamo anche noi, per la parte che ci riguarda, al fatto che comunque abbiamo raggiunto tale risultato. Anche il secondo argomento, oggetto di modifica da parte della Camera,

comportava chiari ed evidenti motivi di incostituzionalità, ma soprattutto uccideva definitivamente piccole e medie aziende, che probabilmente avrebbero chiuso i battenti, mandando a casa decine e decine di persone.

anni, sostenendo che la sanità in quanto tale non può rispondere a motivi di carattere ragionieristico; ci siamo riempiti la bocca tutti quanti con convinzione - alcuni di più ed altri di meno

subiscono - a mio avviso in maniera negativa - il taglio del Ministero dell'economia. Pertanto, richiamiamo tutti i colleghi sia della maggioranza che dell'opposizione che hanno a cuore il tema della salute, il tema del sociale, a fare in modo che prevalga sempre più la logica

Non può dire che ha raggiunto un accordo con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni se poi andiamo a vedere che il protocollo contiene solo vuote e generiche affermazioni sui princìpi di carattere generale, affermazioni non accompagnate da interventi di carattere finanziario.

questi sprechi possano essere attenuati da una verifica attenta e puntuale sugli adempimenti fissati dai piani di rientro ed è quindi importante la disposizione prevista dalla modifica apportata in sede di conversione relativamente alla verifica annuale. Mi auguro - lo dico per la parte della salute al sottosegretario Zucchelli - che la verifica annuale dei piani di rientro

a fare in modo che il tema della salute, che talvolta ha visto scontrare maggioranza ed opposizione su argomenti importanti come quello di dare alle Regioni la possibilità di spendere in maniera seria

Signor Presidente, credo abbia fatto bene il collega Cursi ad evidenziare oggi nel suo intervento

presentammo una serie di emendamenti nei quali si chiedeva proprio di non prevedere

avesse chiesto l'abolizione dei *ticket*. Oggi, grazie al passaggio del decreto dal Senato alla Camera e al suo ritorno, abbiamo visto questa cancellazione. Ma io voglio far riferimento a quanto le Regioni, che saranno beneficiate da questo provvedimento, dovranno, invece, mantenersi attente e scrupolose;

si è intervenuti per ripianare i debiti delle USL prima, delle ASL poi. È sempre intervenuto il Parlamento per dare una mano concreta alla spesa sanitaria. Si disse

delle piccole aziende che operano come fornitori del Servizio sanitario vi è una richiesta impellente di intervento. La giustificazione della Giunta regionale del Lazio è di è di non poter votare la delibera con la quale la Regione dava il via ai pagamenti dei fornitori di beni e servizi del sistema sanitario regionale (debiti fatturati nel 2006 tengo a sottolineare -quindi sotto precise responsabilità della Giunta Marrazzo e dei suoi assessori al bilancio

la manovra di 2 miliardi 554 milioni da parte del Governo e del Parlamento per il decreto "salva *deficit*". Allora i soldi arriveranno. Dobbiamo vedere come poi, caso per caso, le Regioni che ricevono questo denaro possano fare. Allora ho ripreso un intervento in Consiglio regionale di un paio di mesi fa, quando si è aperto un dibattito sulla situazione regionale ed è emerso - guardate caso - che il direttore generale di una grande azienda ospedaliera, il San Camillo-Forlanini - che credo sia ancora la più grande azienda ospedaliera d'Europa

all'ordine dei giornalisti del Lazio e non risultava. Poi ho verificato se fosse stato iscritto in qualsiasi altro ordine dei giornalisti. Invece, scopro che il portavoce del dottor Macchitella, direttore generale dell'azienda San Camillo-Forlanini, è un portantino con la terza media, che riceve lo stipendio di giornalista senza esserlo. Allora, i mezzi arrivano.

dell'ordine del giorno del mondo della cultura e della politica contro la vendita dell'ospedale stesso. Il Forlanini viene venduto per far cassa,

una struttura con una storia ed una tradizione di altissimo livello. Mi dispiace che non sia presente in quest'Aula il presidente della Commissione igiene e sanità, il professor Marino, che conosce quelle situazioni e sa benissimo qual è il livello

allora, come si è verificato in questi giorni, che l'eliambulanza del 118 sia costretta ad uscire dal territorio regionale, per portare i ricoverati in Abruzzo, all'ospedale di Avezzano, perché i posti letto nel territorio della Regione Lazio,

cui devono fare riferimento anche i deputati, i senatori e i dipendenti del Senato e della Camera: si stanno cancellando le strutture ospedaliere e i poliambulatori che hanno convenzione diretta con il Parlamento della Repubblica.

l'opposizione in Consiglio regionale a dire di no al taglio di quel pronto soccorso ma anche un esponente importante della maggioranza ritiene pericoloso tale taglio e la chiusura del pronto soccorso. Per chi non lo quell'ospedale è al centro di un grande quartiere popolare, quale la Garbatella; ma a lor signori questo non importa. Essi tagliano per poi spostare

ASL è davvero al centro del ciclone delle indagini della Polizia giudiziaria per le truffe perpetrate dai dirigenti susseguitisi alla guida di quella azienda.

ma preferiscono perdere un quarto d'ora di macchina. Da Frascati, infatti, basta un quarto d'ora di macchina per recarsi in una struttura d'avanguardia come il Policlinico di Tor Vergata. Il direttore generale di quell'azienda, un altro beneficato un altro beneficato della politica regionale del Lazio, è stato direttore sanitario, poi è andato via, è ritornato, poi è stato il riferimento di alcuni di alcuni importanti Gruppi e di alcuni importanti personaggi della politica; mi dispiace che non ci sia il collega Pasetto che è sempre stato il suo protettore. Ebbene, questo direttore generale si arrabbia

e governano ospedali da 1.300 posti e non sanno nemmeno di cosa si parla nella struttura che governano. Allora ben venga